dopo il 28 settembre, cioè la giornata nella quale il Presidente medesimo riferirà sulla vicenda Telecom alla Camera.

e quindi di affrontare la questione in una successiva seduta, ripeto, dopo il 28 settembre, sulla base di una comunicazione del Presidente del Consiglio. Pertanto, la seduta è da considerarsi

Conferenza dei Capigruppo sarà convocata per decidere il calendario successivo dei lavori dell'Assemblea, praticamente di tutta la settimana.